finestra") *(PD)*. Signora Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli senatrici e senatori, il settore della ricerca continua ad essere nel nostro Paese in una situazione di sofferenza. La spesa per ricerca e sviluppo, che in Italia non raggiunge l'1 per cento del PIL, ci vede ultimi tra i Paesi dell'Unione europea a 15, al di sotto della media dell'Unione europea a 27 ben lontani dal 3 per cento che l'Europa si è data come obiettivo da raggiungere entro il 2010 (e siamo già nel 2009). Anche se consideriamo il rapporto tra cittadini e ricercatori, secondo i dati dell'OCSE per

l'intenzione di rimettere in discussione le procedure di stabilizzazione che erano state previste dalle leggi finanziarie Prodi per il 2007 e per il 2008, procedure che rispondevano all'esigenza di risolvere la drammatica ed annosa situazione dei lavoratori precari. L'orientamento è quello di ostacolare il percorso di risanamento di un'anomala situazione che per anni ha visto l'utilizzazione del lavoro di persone che, in molti casi vincitori o idonei di concorsi o selezioni svolte negli anni passati, non erano e non sono mai state stabilizzate, anche a causa del continuo blocco delle assunzioni. La situazione si presenta drammatica: stiamo infatti parlando di lavoratori - scienziati e personale dei centri di ricerca - altamente qualificati, che per anni hanno svolto con rigore e professionalità il proprio lavoro, per poter dare alla ricerca italiana un ruolo da protagonista anche in ambito internazionale. Per anni migliaia di ricercatori, tecnici, amministrativi hanno lavorato in condizioni difficilissime, garantendo il funzionamento del sistema pubblico della ricerca e dell'università. Il blocco delle procedure di stabilizzazione comporta la dispersione di un patrimonio prezioso costituito da persone, a volte neanche più giovani, che hanno investito la loro vita nella ricerca, magari tornando dall'estero per poter dare il proprio contributo all'Italia, e che vedono svanire la possibilità di avere un futuro lavorativo stabile. L'impossibilità di continuare ad usufruire dei precari storici comporterebbe anche la vanificazione delle risorse ingenti investite nella loro formazione e nei progetti di ricerca e l'aumento, a questo punto inevitabile,

il Governo ha prima riformulato l'emendamento e poi avviato una serie di incontri con i presidenti degli enti di ricerca per l'istituzione di tavoli di confronto. Si tratta però solo di un'apparente soluzione al problema: a quanto mi risulta, mancano i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri autorizzativi per le procedure di stabilizzazione avviate dagli enti di ricerca e non ci sono quindi più i tempi utili per procedere alle ulteriori stabilizzazioni. È quindi realistico pensare che il nuovo termine fissato non sarà sufficiente per procedere non solo alle stabilizzazioni previste con la legge finanziaria 2008, ma neanche a quelle previste con la legge finanziaria 2007. Inoltre, le soluzioni riguardano unicamente i lavoratori con contratto a tempo determinato. Non sembrano esserci invece prospettive per le migliaia di cosiddetti precari invisibili: lavoratori a progetto, contrattisti, borsisti, i quali, se non verranno prese iniziative correttive, vedranno i loro contratti scadere senza possibilità di rinnovo successivamente al 30 luglio di quest'anno. Sono, questi ultimi, vittime di un sistema che non ha indetto concorsi per anni, creando figure precarie, a cui è impedito di avere non solo certezze, ma anche speranze sulle prospettive professionali, speranze che sono indispensabili per poter svolgere il proprio lavoro con l'impegno e anche con la tranquillità psicologica che meriterebbero; quell'impegno, quella tranquillità psicologica che il sottosegretario Pizza insieme a me ha avuto la possibilità, solo una settimana fa, di vedere in tanti ricercatori italiani impegnati, ad esempio, in un'istituzione straniera come il Karolinska Institutet a Stoccolma, in Svezia. Il ministro Brunetta, in un'intervista di qualche tempo fa, affermava che coloro che non saranno assunti, e che quindi perderanno il loro lavoro, «non saranno a spasso, si cercheranno qualcos'altro da fare. La ricerca è questa. I ricercatori sono un po' come capitani di ventura, stabilizzarli è un farli morire». Vorrei ricordare al sottosegretario Pizza, al ministro Brunetta e a tutti i membri del Governo che molti di questi lavoratori hanno alle loro spalle anni di esperienza, spesso anche in altri Paesi. Poter fare esperienza all'estero è senz'altro utile; io stesso a 28 anni ho deciso di continuare i miei studi negli Stati Uniti per coltivare un mio sogno. Ma deve essere una scelta, non si deve essere costretti ad emigrare perché il nostro Paese non offre altre possibilità. È una scelta miope quella di investire nella formazione dei nostri giovani per poi non lasciare loro altra possibilità se non quella di andare all'estero. In questo modo, non solo non riusciremo a trattenere le nostre menti migliori, ma non saremo di attrattiva per nessun ricercatore straniero; una strategia ancor più miope, se consideriamo che oggi viviamo una crisi finanziaria che richiederebbe di investire sul futuro, sui nostri giovani migliori. In un momento come quello che stiamo attraversando, bisognerebbe trovare misure comuni per fronteggiare i problemi di occupazione e sviluppo, puntando sui settori che, nel lungo periodo, possono ridarci fiducia e prospettiva. E invece frustriamo le speranze dei nostri scienziati e rischiamo di paralizzare gli enti di ricerca. I provvedimenti adottati fino a questo momento sono la prova di una visione corta e limitata rispetto ai grandi problemi di questo Paese. Qual è la risposta di programmazione del Governo? L'unica risposta oggi è quella di tagliare i finanziamenti alla ricerca e rendere il settore ancora più precario. La risposta di un Governo che non ha a cuore il settore della ricerca

alle migliaia di precari che stanno lavorando in questi anni con professionalità e dedizione e che potrebbero trovarsi presto senza una posizione. Vi chiedo, inoltre, se non riteniate improcrastinabile aumentare l'investimento sulla ricerca, anche al fine di reagire alla crisi finanziaria in corso e di conseguire gli obiettivi di crescita sanciti nel Consiglio europeo di Lisbona, ritenendo a tal fine indispensabile rafforzare la crescita e l'indipendenza, in particolare, dei ricercatori. Per queste ragioni, ribadendo la mia richiesta di conoscere quali azioni il Governo intenda intraprendere in questo campo, ritengo però necessario imprimere una significativa accelerazione nella direzione di un sistema basato sulla valutazione e sulla valorizzazione del merito, su risorse appropriate e programmate, su un regime fiscale incentivante Grazie Proprio in merito a questi specifici obiettivi, mi auguro quindi che in futuro ci sia una necessaria e più adeguata riflessione nell'attività parlamentare e di Governo. PRESIDENTE. Il rappresentante

del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, alcuni quesiti che attengono agli effetti che determinerà nell'ambito degli enti di ricerca la disposizione generale di riordino della disciplina sulla stabilizzazione, contenuta nell'articolo 7 del disegno di legge di cui all'Atto Senato n. 1167, recante «Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali». Preliminarmente si fa presente che gli enti di ricerca, aventi per l'anno 2008, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, risorse finanziarie disponibili per le assunzioni, comprese le stabilizzazioni, hanno presentato regolare richiesta di autorizzazione alle assunzioni. Il Dipartimento della funzione pubblica ha provveduto, prima della predisposizione dei relativi provvedimenti, a concludere le preliminari procedure istruttorie, come previsto dalla norma, a predisporre i prescritti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ad inoltrare gli stessi, già firmati dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al Ministero dell'economia e delle finanze per acquisire il concerto e quindi la firma del relativo Ministro. La trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze è avvenuta, per tutti i predetti schemi di provvedimento, prima del 31 dicembre scorso. Si segnala che il suddetto Dipartimento ha riconsiderato, a fine anno 2008, l'istruttoria sulle richieste pervenute, alla luce delle novità introdotte dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 novembre 2008 n. 180, convertito in legge dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, che, nel recare disposizioni urgenti "per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca", ha previsto di escludere gli enti di ricerca dalla riduzione, non inferiore al dieci per cento, della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico del personale non dirigenziale,

Quest'ultima novità legislativa, infatti, ha fatto venir meno in capo ai predetti enti l'obbligo di ridurre le dotazioni organiche e quindi ha comportato in molte circostanze la riproposizione da parte degli stessi di nuove richieste di assunzione per l'anno 2008, alla luce del nuovo quadro normativo. Si ricorda, sempre per quanto riguarda le autorizzazioni ad assumere per l'anno 2008, che il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, è intervenuto per dettare alcune disposizioni di proroga. In particolare, l'articolo 41, comma 1, prevede, anche per codesti enti, che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, è prorogato al 31 dicembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009.

potranno essere effettuate entro il termine massimo del 31 dicembre 2009. Per quanto riguarda le assunzioni relative all'anno 2009, è in corso di emanazione la circolare che detta le istruzioni per procedere alle prescritte autorizzazioni. Le previsioni fanno ritenere possibile l'adozione dei relativi provvedimenti entro il primo semestre dell'anno e, conseguentemente, le assunzioni ed eventuali stabilizzazioni potranno concludersi nei tempi con l'utilizzo delle risorse che il legislatore ha stanziato per l'anno 2009. A tale proposito è necessario precisare che le disposizioni in materia di stabilizzazione negli enti di ricerca, contenute nelle leggi finanziarie 2007 e 2008, stanziavano risorse per dette finalità solo per gli anni 2007, 2008 e 2009, prevedendo che la relativa procedura speciale di reclutamento potesse svolgersi solo fino al 2009

recato dall'articolo 7 dell'Atto Senato n. 1167, mira a definire gli effetti del percorso avviato con la precedente legislatura, introducendo la possibilità per il triennio 2009-2011 di procedure concorsuali speciali, volte a valorizzare l'esperienza professionale in particolare della platea di soggetti non stabilizzati o a causa del venir meno, dopo il 2009, di risorse finanziarie da destinare alle relative assunzioni o perché, comunque, non rientranti nel fabbisogno di personale dell'ente. Come rilevato nell'interpellanza, è vero che l'avvio delle predette procedure concorsuali è subordinato all'effettivo fabbisogno degli enti, al superamento delle prove da parte dei candidati che possono usufruire della riserva, alla disponibilità di risorse finanziarie per l'assunzione. Non sussiste certezza, quindi, in merito all'effettiva assunzione dei soggetti interessati. La circostanza descritta non è tuttavia molto diversa da chi partecipa ad un concorso, magari senza godere di posti riservati e, pur risultando vincitore, non può essere assunto a causa dei vincoli assunzionali che riguardano le amministrazioni pubbliche. La giurisprudenza si è più volte espressa ritenendo detti soggetti titolari di un interesse legittimo all'assunzione e non di un diritto soggettivo. Per quanto riguarda il fatto di anticipare, con la norma *in itinere*, gli effetti della conclusione delle procedure di stabilizzazione al 30 giugno 2009, si ritiene che ciò non precluda, agli enti di ricerca, di utilizzare, per l'anno in corso, i finanziamenti previsti per le connesse assunzioni, considerato appunto che il Dipartimento per la funzione pubblica provvederà, come detto, ad adottare per tempo i relativi provvedimenti di autorizzazione ad assumere. Circa i soggetti in possesso dei prescritti requisiti per la stabilizzazione, è utile segnalare che il numero si aggira intorno alle 2.000 unità, come riscontrato a seguito di un monitoraggio mirato fatto con gli enti di ricerca, e non alle 60.000 come riferito dagli interpellanti. Sotto il profilo generale, si sottolinea che la ricerca è uno di quei settori caratterizzati da evoluzioni continue che non si conciliano con un fabbisogno ordinario, costante e continuativo, delle stesse professionalità. I ricercatori, infatti, vengono utilizzati in stretta connessione con il finanziamento dei progetti connessi agli obiettivi di sviluppo perseguiti, tenuto conto dei programmi di ricerca nazionali e di quelli comunitari ed internazionali. In detto settore, in sostanza, l'utilizzo di tipologie di lavoro flessibile è in linea con le esigenze istituzionali degli enti e con le caratteristiche delle attività svolte che sono destinate ad avere una durata limitata nel tempo in ragione del progetto e delle risorse assegnate. Risulterebbe, perciò, privo di utilità per gli enti e contrario ai principi di economicità, assumere a tempo indeterminato tutto il personale utilizzato per ricerche di durata prestabilita. Secondo le regole a rilevanza costituzionale vigenti in materia di accesso al pubblico impiego, anche il reclutamento a tempo determinato avviene per pubblico concorso. Il tempo determinato trova il suo presupposto in attività che non rientrano, come detto, nel fabbisogno ordinario dell'ente. deve, infatti, tenere conto che per quest'ultimo fabbisogno occorre bandire solo procedure concorsuali a tempo indeterminato. Il corretto utilizzo della medesima programmazione del fabbisogno e delle scelte di reclutamento operate risulta anche coerente con il diverso affidamento dei partecipanti e dei non partecipanti al bando di concorso per l'assunzione a tempo determinato. In relazione a detto affidamento non può, nel tempo, trasformarsi il reclutamento per il tempo determinato in una modalità di accesso a tempo indeterminato, al di là della natura pubblica della procedura. Ciò, infatti, striderebbe con il regolare, trasparente e corretto funzionamento del sistema, inficiando l'attività amministrativa di mancato rispetto delle regole di imparzialità. Si ritiene, pertanto, che la soluzione prospettata dall'articolo 7 dell'Atto Senato n. 1167 sia quella che meglio contempera i principi inderogabili dell'ordinamento giuridico con l'esigenza di riconoscere un valore all'esperienza professionale maturata dai soggetti che hanno maturato l'anzianità di servizio prescritta. Inoltre, la possibilità di mantenere in piedi i contratti di lavoro flessibile del suddetto personale, eventualmente anche in deroga alla normativa vigente in materia, sarà opportunamente valutata dopo il monitoraggio indicato nel citato articolo sulla base dei criteri forniti dal decreto del Presidente del Con riferimento alle ulteriori richieste, il Governo ritiene sicuramente improcrastinabile l'investimento sulla ricerca e, a conferma della necessità e dell'urgenza di un approccio innovativo nei confronti soprattutto dei giovani ricercatori, già con il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, ha provveduto a modificare le procedure di reclutamento degli stessi, relativamente alla composizione delle commissioni dei concorsi e alla valutazione dei candidati, secondo criteri e parametri riconosciuti anche in ambito internazionale; è stata anche prevista la chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero da almeno un triennio, che ricoprano una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie e che abbiano conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne è chiesto il rientro. Lo stesso provvedimento, inoltre, allo scopo di valorizzare il merito dell'attività di ricerca svolta, dal 1° gennaio 2011 ha previsto, sempre per i ricercatori, scatti biennali previo accertamento, da parte dell'autorità accademica, dell'effettuazione nel biennio precedente di pubblicazioni scientifiche. È stata data anche attuazione all'articolo 4-*bis*, comma 17, del decreto-legge 3 giugno 2008, 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, disponendo assegnazioni agli enti di ricerca vigilati, finalizzate al reclutamento aggiuntivo di ricercatori per complessivi 517 posti, da coprire con le risorse stanziate per l'anno 2008, pari a 30 milioni di euro a regime, che non necessitano di autorizzazioni da parte della Funzione pubblica. Il Ministero, nella consapevolezza della necessità di favorire concretamente il ricambio generazionale all'interno degli atenei e degli enti di ricerca pubblici destinando adeguate risorse al finanziamento di progetti di ricerca coordinati da giovani ricercatori non strutturati, e nella considerazione dell'esigenza concreta di selezioni meritocratiche, basate sull'effettiva eccellenza scientifica, misurata sul campo e connessa anche con la gestione ed il coordinamento di progetti di ricerca a rete (*community network*), che consenta di superare i tradizionali limiti della frammentazione disciplinare, con il decreto direttoriale 19 dicembre 2008 ha emanato il bando FIRB (Fondo per

non ancora strutturati presso gli atenei italiani, statali o non statali, e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR; per la linea d'intervento 2, a giovani docenti o ricercatori, di età non superiore a 38 anni, già strutturati presso le medesime istituzioni. Il programma si concretizza nella presentazione, da parte dei soggetti di cui alle linee d'intervento predette, in qualità di responsabili di progetto e secondo le modalità e nei termini indicati, di progetti di ricerca fondamentale, anche a rete, di durata almeno triennale. La valutazione scientifica dei progetti, ai fini dell'eventuale finanziamento ministeriale, è effettuata separatamente per ciascuna linea di intervento da una specifica commissione di esperti, anche di nazionalità non italiana, nominata dal Ministero su proposta della commissione di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, sia mediante valutazione della documentazione presentata, sia mediante apposite audizioni. Per i giovani dottori di ricerca di cui alla linea d'intervento 1, l'ammissione al finanziamento comporta, a pena di decadenza, il conferimento, da parte delle istituzioni partecipanti alla sperimentazione, di appositi contratti di durata almeno triennale, ai sensi della normativa vigente. Al termine dei progetti, una commissione di esperti di settore, anche di nazionalità non italiana, procederà ad una valutazione *ex post* incentrata sulle attività svolte e sui risultati conseguiti, fornendo un giudizio complessivo e conclusivo. Anche il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha provveduto, in data 29 dicembre 2008, ad impegnare tutte le somme del finanziamento previsto per l'anno 2008, relative ai programmi della ricerca sanitaria. Nella medesima data sono stati anche pubblicati i bandi per la ricerca finalizzata, per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la sicurezza alimentare ed il bando per i ricercatori di età inferiore ai 40 anni: i quattro bandi sono consultabili, da tale data, sul sito Internet del Ministero, "Settore Salute". Per quanto riguarda le erogazioni liberali, il nostro sistema tributario già prevede una serie di agevolazioni fiscali, nella forma di detrazioni d'imposta e di deduzioni, per i soggetti che effettuano erogazioni liberali in favore di organizzazioni che svolgono ricerca scientifica.

che prevede l'integrale deducibilità dal reddito, per i soggetti passivi IRES, dei fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, in favore di università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici,

che prevede la deducibilità, nel limite del 10 per cento del reddito e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui, delle liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'IRES in favore di fondazioni e associazioni riconosciute, che svolgono o promuovono ricerca scientifica. Tale deduzione non può cumularsi con ogni altra agevolazione prevista, a titolo di deduzione o di detrazione, da altre disposizioni di legge.

l'articolo 15, comma 1, del TUIR, che per i soggetti IRPEF prevede, alla lettera *h)*, una detrazione dall'imposta lorda, nella misura del 19 per cento, delle erogazioni in denaro a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti territoriali, di enti ed ed istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute, senza scopo di lucro, aventi per oggetto l'attività ovvero la promozione delle attività

fatte a favore di persone giuridiche che perseguono finalità di ricerca scientifica, per un ammontare non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato. L'attuale L'attuale sistema delle agevolazioni fiscali sembra essere un adeguato sostegno alla ricerca scientifica ed un sufficiente incentivo alle erogazioni liberali effettuate in favore della stessa. Un eventuale ampliamento ed allargamento delle agevolazioni fiscali potrebbe essere valutato soltanto in una situazione economica più favorevole.

onorevoli senatrici e senatori, posso ritenermi parzialmente soddisfatto per alcuni aspetti tecnici che il Sottosegretario ha fornito oggi all'Aula; in particolare, il termine per la stabilizzazione dei precari della ricerca sia stato spostato al 31 dicembre 2009. Ciò può far sperare che molti di questi dipendenti di enti pubblici impegnati in ricerca possano in effetti vedere riconosciuto il lavoro che hanno svolto negli anni. Debbo però dichiararmi insoddisfatto per l'impostazione generale degli investimenti in ricerca. Farò alcuni commenti di carattere generale e altri specifici su due bandi che il Sottosegretario ha citato e che conosco molto bene, nei dettagli.

alcuni milioni di abitanti in più, come la Germania e la Francia, hanno rispettivamente 280.000 e 210.000 persone impegnate in ricerca. Quello che però a me preoccupa maggiormente è quanto viene investito e quanto viene indirizzato alle menti più giovani. Forse è un numero che non è noto a tutti

anni. Credo che questi siano numeri molto chiari che debbono farci capire come è diversa la nostra situazione. Cito altre due decisioni importanti di Governi dell'Unione europea. Il Governo Sarkozy, a ottobre, in pieno crollo di Wall Street, ha deciso

Il Governo svedese, che è già il primo in Europa con il 4,27 per cento del PIL investito in ricerca, ha deciso urgentemente, nelle ultime settimane, di investire altri 500 milioni di corone in ricerca. Noi eravamo all'1,1

l'onorevole senatrice interrogante, prendendo spunto dalla realtà di Torino, pone in via generale il tema della concentrazione degli alunni stranieri in alcuni territori e in alcune scuole o classi, soffermandosi, in particolare, sull'esigenza dell'apprendimento della lingua italiana come seconda lingua da parte degli alunni non italofoni. Come è noto, sul tema dell'integrazione degli alunni stranieri il Governo ha recentemente riferito sia alla Camera, il 9 e il 14 ottobre 2008, sia in questa stessa sede, il 18 dicembre scorso, in relazione a varie mozioni al riguardo presentate. Nel confermare quanto già riferito nelle suddette sedi, faccio presente che nella circolare ministeriale n. 4 del 15 gennaio 2009, relativa alle iscrizioni degli alunni per il prossimo anno scolastico, una specifica attenzione è stata dedicata proprio alle iscrizioni degli alunni con cittadinanza non italiana, in considerazione del carattere strutturale e della complessità che il fenomeno di alunni con cittadinanza non italiana ha assunto da tempo. Nella suddetta circolare è stato richiamato il quadro normativo attualmente vigente ed in particolare l'articolo 45 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999. Per ciò che riguarda specificamente la rilevata esigenza di evitare la concentrazione di alunni con cittadinanza non italiana e i conseguenti squilibri e disagi, nella citata circolare è stata sottolineata l'opportunità che le istituzioni scolastiche realizzino accordi di rete per una razionale distribuzione territoriale delle domande, procedendo, quindi, ad un'equa assegnazione degli alunni alle diverse classi. A tal proposito, è stata evidenziata l'esigenza che i direttori generali degli uffici scolastici regionali promuovano le iniziative ritenute più opportune per l'attivazione degli accordi di rete. Sono state inoltre fornite indicazioni affinché le istituzioni scolastiche, possibilmente con azioni in rete, sollecitino o assecondino attivamente le iniziative degli enti locali e/o di altri soggetti a livelli istituzionali per l'adozione di misure di prevenzione, orientamento e controllo circa l'assolvimento dell'obbligo di istruzione ed è stata pure sottolineata la necessità che nelle città e nei grandi centri urbani, in cui sono presenti ampie reti di scuole, le iscrizioni di alunni con cittadinanza non italiana siano gestite in maniera partecipata e programmata, in modo che la domanda e l'offerta di servizi scolastici risultino equamente distribuite. È stata anche sottolineata l'opportunità che, nella predisposizione degli accordi, siano previste intese con gli enti locali per favorire l'attivazione di misure di accompagnamento, (trasporti, mense, e così via) utili al conseguimento di un'equilibrata distribuzione della domanda, nonché intese con associazioni del volontariato e del privato sociale per specifiche azioni di integrazione. infine, sottolineata la fondamentale importanza dell'instaurazione di un attento e proficuo rapporto tra le scuole e le famiglie dei minori iscritti, eventualmente facilitato dall'intervento di mediatori culturali e di operatori del volontariato sociale e di associazioni interculturali. Quanto poi alla richiesta di interventi per favorire l'apprendimento della lingua italiana, tale esigenza è stata rilevata in più punti della suddetta circolare. In particolare,

Grazie che l'assegnazione definitiva alla classe sia preceduta da una fase di alfabetizzazione strumentale e di conoscenza linguistica, anche all'interno di specifici gruppi temporanei di apprendimento, finalizzata a favorire un efficace e produttivo inserimento, utilizzando le eventuali ulteriori disponibilità dell'organico dì istituto. È stata, inoltre, fornita indicazione affinché le istituzioni scolastiche, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, favoriscano iniziative volte a migliorare la conoscenza e l'apprendimento della lingua italiana e a diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza. Sono state pure ricordate, infine, le possibilità in proposito offerte dai corsi di alfabetizzazione per adulti, previsti dal decreto ministeriale del 25 ottobre 2007. In merito poi alla richiesta volta a conoscere le risorse che si intendono destinare all'insegnamento della lingua italiana come seconda lingua per gli studenti di recente immigrazione, ricordo che esiste il programma denominato «Scuole aperte». Detto programma, confermato per il corrente anno scolastico, prevede quattro aree tematiche oggetto di finanziamenti, tra cui quella relativa proprio al piano di insegnamento di italiano L2. Le risorse finanziarie ad esso dedicate ammontano a 4.500.000 euro e vengono ripartite tra gli uffici scolastici regionali e provinciali proprio in base alla presenza di alunni di recente immigrazione delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Questo finanziamento si pone in continuità e a sostanziale integrazione delle iniziative progettuali realizzate dalle singole istituzioni autonome con i fondi previsti all'articolo 9 del contratto quali misure incentivanti per le aree a rischio e a forte processo immigratorio. Detto questo in via generale, per quel che si riferisce specificamente alla situazione della città di Torino, la direzione scolastica regionale per il Piemonte ha fornito dettagliati elementi di conoscenza sia in ordine ai dati di carattere statistico, sia in ordine alle numerose iniziative attuate nel territorio dalle reti di scuole sulla base di progetti per l'insegnamento di italiano seconda lingua rivolti e ai neo-arrivati e, per facilitarne lo studio, agli allievi di seconda generazione. Dai dati statistici forniti dalla stessa direzione scolastica regionale, risulta l'obiettiva difficoltà di porre il limite massimo del 10 per cento di allievi stranieri per classe, cui tenderebbe invece la mozione menzionata nell'atto in discussione, in considerazione che tale limite, per molti quartieri di Torino, è ampiamente al di sotto della media.

della prima infanzia e materna (neppure di quella primaria di primo e secondo grado). Ringrazio pertanto il Sottosegretario per aver dilatato la sua osservazione più complessivamente all'inserimento degli alunni stranieri in ogni ordine di scuola, però l'interrogazione muoveva dalla richiesta

dall'articolato commento che il Sottosegretario ha fatto della circolare ministeriale del gennaio 2009 sull'inserimento degli stranieri nelle scuole devo dedurre che quella richiesta è stata respinta,

sul fatto che debba essere l'autonomia della rete delle scuole, insieme agli enti locali, a trovare il giusto livello d'integrazione e che debba essere inoltre riconfermato quel fondo di 4 milioni, di cui all'articolo 9 del Ora, se le cose stanno così, notando il fatto politico e culturale del rifiuto di una proposta durissima che veniva applicata esplicitamente alle scuole dell'infanzia, prendo atto del fatto che ripercorriamo passi già fatti, vale a dire l'autonomia scolastica, l'integrazione e, aggiungerei, l'evoluzione della popolazione scolastica tra gli stranieri di prima e di seconda generazione. Infatti, un conto

apprezzamento anche degli uffici scolastici regionali, particolarmente per quello della mia Regione, che conferma il *budget* di 600.000 euro per questo punto dell'articolo 9 del contratto nazionale di lavoro.

dopo i tagli dolorosamente subiti con l'ultima finanziaria e gli ultimi provvedimenti e verificare se queste linee di azione e culturali, che io apprezzo, potranno o non potranno essere concretamente riconfermate.

con riferimento all'interrogazione del senatore Lumia, si fa presente che la legge n. 279 del 2002, che ha riformato l'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, ha conferito ai detenuti sottoposti al regime speciale strumenti completi di impugnazione avverso il provvedimento ministeriale che ne determina l'applicazione, individuando competenze, funzioni e poteri dei giudici chiamati a sindacare la legittimità dei decreti applicativi del regime in questione. Infatti, subito dopo l'entrata in vigore della nuova legge e in conseguenza della effettività della tutela giurisdizionale garantita dalla normativa, si è registrato un forte incremento dei ricorsi e, parallelamente, una maggiore incidenza degli annullamenti dei decreti ministeriali. Il dato relativo alle declaratorie di inefficacia pronunciate dai tribunali di sorveglianza va dunque letto parallelamente a questa incisiva crescita del numero dei reclami presentati. Tali annullamenti, in alcuni casi, hanno riguardato gli storici *boss* della criminalità organizzata, rispetto ai quali il consistente numero di anni trascorso in stato di carcerazione è stato valutato dall'autorità giudiziaria come elemento da cui desumere il venir meno dell'attualità del collegamento con l'associazione malavitosa di appartenenza. Di fatto, quindi, la corretta gestione dello strumento penitenziario del regime speciale dell'articolo il conseguente raggiungimento delle finalità preventive cui lo stesso risulta preordinato ha finito, talvolta, per essere utilizzato *a contrariis*, come argomentazione per sostenere il venir meno dei presupposti legittimanti la protrazione dell'applicazione del regime suddetto. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, al fine di contrastare alcune impostazioni giurisprudenziali che avevano condotto all'annullamento di un certo numero di provvedimenti di applicazione, ha cercato di intervenire su diverse linee. In prima battuta, ha argomentato in modo specifico sui punti oggetto di disputa interpretativa, predisponendo articolate argomentazioni giuridiche da mettere a disposizione delle autorità giudiziarie competenti alle impugnazioni. L'amministrazione penitenziaria si è poi adoperata per creare un rapporto di fattiva collaborazione con la Direzione nazionale antimafia, in modo da elaborare linee interpretative comuni, volte ad agevolare l'attività degli organismi chiamati a proporre le impugnazioni. È stato adottato, infatti, un modulo organizzativo che consentisse di comunicare tempestivamente alla Direzione nazionale antimafia la presentazione del ricorso e la data dell'udienza per la sua discussione.

In esito a tali iniziative e sulla base dei ricorsi dei procuratori generali così provocati, la Cassazione ha preso posizione sulle questioni controverse e, nell'accogliere la tesi ministeriale, ha di fatto cercato di correggere l'impostazione originariamente assunta da alcuni tribunali di sorveglianza. Tanto premesso, si segnala che l'attività di impugnazione da parte dei procuratori generali si è sviluppata a partire dall'anno 2003 e costituisce, perciò, una novità prodotta dallo sforzo congiunto di Direzione nazionale antimafia e Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria: in assenza di tale iniziativa di stimolo, la stessa si sarebbe tradotta in una facoltà soltanto teorica e l'intero sistema del regime speciale di detenzione sarebbe inesorabilmente franato.

rilevanti da portare a sostegno dei provvedimenti di proroga costituisce, quindi, la principale risorsa per consentire un'adozione certa e durevole del provvedimento ministeriale. L'amministrazione, infatti, si è impegnata ad adottare un modello di decreto che coniughi il quadro generale della funzione preventiva dell'istituto con gli elementi ricavati dalla posizione individuale del detenuto, così da rafforzare gli aspetti che presentano una maggiore vulnerabilità rispetto agli interventi dell'autorità giudiziaria. Inoltre, d'intesa con le magistrature requirenti, sono stati poi riproposti, ove possibile, i decreti di 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario per alcuni soggetti di elevata caratura criminale che, su provvedimento dei competenti tribunali di sorveglianza, erano stati reimmessi nei circuiti ordinari. Al fine di rendere più efficace e consistente la finalità preventiva propria del regime speciale e scongiurare il pericolo che gli esponenti della criminalità organizzata siano in grado di continuare a determinare le strategie dell'organizzazione di riferimento, con nota del 19 luglio 2008 indirizzata a tutti gli istituti dotati di sezione 41-*bis*, sono state ribadite e sottolineate le disposizioni contenute nella circolare dipartimentale del 9 ottobre 2003, relativa alla concreta attuazione del regime detentivo speciale. A tal proposito, le direzioni dei citati istituti sono state sollecitate ad attenersi in maniera assoluta, senza deroghe od eccezioni, alle limitazioni contenute nella circolare e nel decreto applicativo, utilizzando, necessario in maniera rigida e costante, gli strumenti e gli interventi, anche di carattere strutturale, che l'ordinamento penitenziario mette a disposizione per evitare comunicazioni tra ambienti penitenziari diversi. È stato, inoltre, vietato l'ingresso, nei reparti di 41-*bis* a soggetti diversi dal personale di servizio appositamente individuato. Con riferimento, poi, alla ipotizzata necessità di disporre visite ispettive presso i tribunali di sorveglianza, si deve osservare la mancata indicazione, da parte dell'onorevole interrogante, di specifiche anomalie verificatesi in relazione alle revoche disposte dai tribunali in parola, fa ritenere che l'adozione dei provvedimenti in questione sia da ricollegare al fisiologico svolgimento dell'attività giurisdizionale di competenza degli uffici. Eventuali critiche, mosse ai singoli provvedimenti adottati, dovranno essere fatte valere, pertanto, nelle competenti sedi deputate al vaglio giurisdizionale di tali atti, atteso che non ne viene denunciata l'abnormità o la manifesta contrarietà a disposizioni di legge, cui consegue l'iniziativa di carattere disciplinare. Per quanto riguarda, invece, gli interventi legislativi in materia di 41-*bis*, si segnala la presentazione, nell'ambito del disegno di legge n. 733 di iniziativa governativa recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di un emendamento finalizzato alla modifica del regime di carcere duro previsto dall'articolo 41-*bis*.

«per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso». È stato previsto, inoltre, che il provvedimento di sospensione abbia durata pari a quattro anni e sia prorogabile per successivi periodi, ciascuno pari a due anni (laddove, attualmente, la norma dispone che il provvedimento abbia durata non inferiore ad un anno e non superiore a due e che la proroga sia pari ad un anno). È rimasto fermo il principio secondo il quale la proroga potrà essere disposta soltanto quando risulti che non sia venuta meno la capacità del detenuto di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva, ma si è voluto specificare che il mero decorso del tempo non costituirà, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o per dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa. Si sottolinea, inoltre, che i detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione saranno ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, ovvero in sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e custoditi custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria. È stato previsto, infine, che dalla sospensione delle normali regole di trattamento derivino automaticamente alcune conseguenze ulteriori, quali la limitazione ad un unico colloquio mensile (peraltro sottoposto a controllo auditivo, registrazione e videoregistrazione) e la limitazione della permanenza all'aperto in gruppi di quattro persone e per due ore al giorno, onde assicurare l'assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità. Sotto il profilo processuale, è stato disposto che la competenza a decidere sul reclamo presentato dal detenuto o dal suo difensore avverso il provvedimento di applicazione o di proroga di sospensione delle normali regole di trattamento, spetti sempre al tribunale di sorveglianza di Roma e non più a quello avente giurisdizione sull'istituto nel quale il sottoposto al regime di carcere duro era recluso al momento della prima applicazione. Tale ultima previsione è stata inserita proprio al fine di risolvere le difficoltà derivanti dall'interpretazione, non sempre uniforme, operata dai diversi tribunali sull'articolo 41-*bis*. Con le modifiche enunciate si è cercato, in buona sostanza, di ripristinare l'originario rigore del regime detentivo speciale, al fine di rendere sempre più difficile per i detenuti e, in particolare per i condannati per associazione mafiosa, i collegamenti con i gruppi criminali di appartenenza.

di ripristino del regime di carcere duro firmati dal Ministro della giustizia il 29 luglio 2008 nei confronti del boss Nino Madonia e il 14 gennaio ultimo scorso nei confronti del boss Domenico Ganci. In entrambi i casi risulta evidente l'attività di completo raccordo e di stretta collaborazione intercorsa tra il Ministro della giustizia, il Dipartimento dell'amministrazione giudiziaria e la direzione distrettuale antimafia di Palermo, Palermo, che ha permesso in tempi estremamente ristretti di dimostrare la reale pericolosità di entrambi i detenuti e la loro capacità attuale di mantenere collegamenti con l'esterno e con le organizzazioni malavitose di appartenenza.

mi convince la prima parte del suo ragionamento in cui ha fatto un'analisi descrittiva dei problemi che l'articolo 41-*bis* ha incontrato in questi ultimi anni mi convince anche l'apprezzamento nei confronti del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per il lavoro svolto nel tentativo di bloccare un'interpretazione sbagliata che si è data della normativa riferita al 41-*bis* e per le misure concrete che sono state poste in essere.

Sottosegretario Caliendo, la dimensione ispettiva non manca a questo Ministero, né manca all'attuale Ministro. Le cronache giudiziarie del nostro Paese sono piene di di una solerte capacità del Ministero d'intervenire ogni volta che si aprono, spesso a mio avviso in modo errato, questioni interne all'attività giudiziaria. Spesso si è troppo solerti e si dà addirittura l'impressione che l'attività ispettiva sia esercitata per mortificare

l'azione penale nell'esercizio della giurisdizione, nel rispetto dell'altro grande principio dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. Sui tribunali di sorveglianza un'attività Eppure molti di essi, come è stato accertato in passato nella stessa Commissione parlamentare antimafia, hanno in modo evidente forzato l'interpretazione della legge:

come sempre avviene, comunicare con l'esterno e garantire una linea di comando interno che ha fatto tanti danni, perché così si stabilisce chi deve pagare il pizzo, quale appalto truccare

Grazie si rappresenta che la manifestazione Festival dei Due Mondi si è regolarmente svolta, come tutti gli anni, nel periodo estivo e sempre nella sede storica di Spoleto. Tutto ciò nonostante un contenzioso insorto tra la Fondazione Festival dei Due Mondi e l'Associazione Festival dei Due Mondi, quest'ultima finanziata dal Ministero per i beni e le attività culturali fino all'anno 2007. Infatti nel 2008, considerato che lo statuto impone alla Fondazione di assicurare la continuità alla manifestazione spoletina, la Fondazione stessa ha provveduto direttamente alla realizzazione dell'evento in considerazione delle difficoltà economiche in cui versava l'Associazione. Pertanto, il Ministero non ha preso in considerazione la domanda di contributo presentata dall'Associazione, essendo carente dei requisiti sostanziali prescritti dalla normativa vigente; in particolare l'istanza non era corredata da un preventivo artistico dei concerti previsti. Il Ministero, invece, proprio allo scopo di dare continuità al Festival dei due mondi, ha accolto la richiesta di finanziamento presentata dalla Fondazione, il cui direttore artistico è Giorgio Ferrara, ed allo stesso organismo ha assegnato il contributo finalizzato alla realizzazione dell'evento in argomento. Infine, si porta a conoscenza della senatrice Spadoni Urbani che l'importo complessivo del contributo assegnato dallo Stato per le attività musicali spoletine per l'anno 2007 è stato di 1 milione di euro, mentre per il 2008 è stato portato a 1.235.000 euro. Il Ministro, e il Sottosegretario che vi parla, è comunque disponibile ad accettare proposte ed iniziative condivise per sostenere, anche meglio del passato, questa iniziativa che dà lustro non solo all'Italia ma al mondo intero.

le risorse che sono state messe in campo, il risultato dell'evento, che ha avuto, per alcuni, una buona eco, mentre per altri meno, nonché le problematiche che dopo l'evento - come anche prima - sono rimaste e permangono.

perché con l'evento si crea la comunicazione. Sappiamo come vanno le cose: nessuno investe se non c'è un ritorno. Mi auguro, sottosegretario Giro, che lei voglia, insieme al Ministro, che è sempre stato sensibile a questi problemi, pensare che Spoleto e il suo Festival sono estremamente importanti come evento culturale per il Paese e per quella collettività. L'Umbria ha bisogno del Festival dei Due Mondi. Spoleto, che è stata trasformata da città industriale, postindustriale, a città culla della cultura per l'Umbria, ha bisogno di attenzione, sia in termini di risorse sia, e soprattutto, in termini di interesse e di promozione da parte di questo Governo.

con riferimento all'interrogazione della senatrice Vicari relativa all'Archivio storico multimediale del Mediterraneo, occorre ripercorrere, brevemente, i passaggi più importanti riguardanti lo sviluppo del progetto. Realizzato dall'Archivio di Stato di Catania, il progetto, che costituisce una importante innovazione nel panorama delle iniziative di diffusione *on line* delle conoscenze e delle fonti storiche, propone e promuove la rilettura della storia del Mediterraneo del secondo millennio attraverso una vastissima mole di documenti e di collezioni cartografiche conservati negli archivi storici dell'Italia e dei Paesi del Mediterraneo. Essi, opportunamente digitalizzati, schedati e organizzati come banca dati in un unico archivio multimediale, vengono resi fruibili *on line* attraverso un portale multilingue dotato di innovative funzioni di ricerca. L'immenso patrimonio documentale confluito nella banca dati sarà consultabile mediante un'interfaccia disponibile in sei lingue (italiano, francese, spagnolo, inglese, arabo, ebraico), requisito, quest'ultimo, che corrisponde al respiro internazionale dell'iniziativa e ne facilita l'ulteriore sviluppo tra i Paesi che vi aderiscono. La prima fase del progetto, già finanziata dal CIPE con 7 milioni di euro (delibera CIPE 17/2003), si è conclusa dopo circa due anni e mezzo di lavoro (metà 2006-fine nel pieno rispetto dei tempi progettuali e contrattuali. Complessivamente è stata costituita una banca-dati iniziale di circa 350.000 immagini ad alta risoluzione, corredate da 62.000 schede catalografiche. In merito alle specifiche domande poste dalla senatrice Vicari, si evidenzia: 1) l'iniziativa ha avuto positivi effetti occupazionali. Infatti, il Raggruppamento temporaneo d'imprese, con il Consorzio Engineering S.p.a Grazie per la gestione della rete e dell'hardware: 3 esperti di sistema; per la realizzazione del portale: 7 analisti e programmatori; per la schedatura e digitalizzazione del materiale: 14 coordinatori, 44 schedatori e 13 tecnici della digitalizzazione; per la traduzione dei regesti: 2 coordinatori e 20 traduttori; per la redazione del portale: 3 unità di personale di redazione); il progetto è stato rimodulato nel 2007 allo scopo di implementare la banca-dati mediante 2.000 descrizioni in regesto (breve riassunto) 3) la mancata adesione dell'Archivio di Stato di Palermo consegue alla situazione logistica delle sedi, in corso di ristrutturazione. Tuttavia, è intendimento del Ministero disporre tutte le opportune iniziative per far sì che sia l'Archivio di Stato di Palermo, sia qualche altro importante istituto, contribuisca all'arricchimento della banca dati dell'Archivio storico multimediale con l'inserimento dei più significativi documenti medievali coerenti con lo spirito e la vocazione mediterranea del progetto; 4) il Ministero, che attribuisce grandissimo rilievo all'iniziativa, anche in considerazione della sua integrazione nel Sistema archivistico nazionale, provvederà a richiedere ulteriori fondi al CIPE per consentire l'implementazione della banca-dati con la documentazione dell'età moderna e contemporanea, selezionando quei percorsi di ricerca che individuino la pluralità dei Paesi del Mediterraneo come entità unitaria e integrata in una rete di rapporti culturali e socio-economici; 5) il Ministero ritiene inoltre necessaria una ulteriore internazionalizzazione del progetto, attraverso la promozione delle caratteristiche tecniche del portale e degli strumenti disponibili per l'integrazione con i diversi sistemi archivistici nazionali dei principali Paesi dell'area del Mediterraneo; del Mediterraneo; 6) infine, in considerazione del fatto che il progetto è stato interamente realizzato, sarà cura di questo Ministero organizzare una presentazione all'opinione pubblica e agli esperti, non soltanto come momento di verifica dell'attività svolta ma anche come importante occasione di promozione e di valorizzazione culturale e scientifica

alla presentazione di tutto il lavoro svolto in questi anni dal Ministero, che potrebbe essere anche motivo di richiesta di implementazione di ulteriori fondi per aprire anche ad altri Paesi che sono interessati a questo processo. È inutile ripetere l'importanza di tutto ciò, soprattutto in un'ottica di pace e di cooperazione con i Paesi del Mediterraneo. È inutile sottolineare come la Sicilia sia la terra più idonea ad essere capofila del Mediterraneo. Proprio per queste considerazioni, l'unico punto del quale non sono soddisfatta per quello che è stato fino ad

a questa fase. Mi rendo conto che i motivi possono essere tanti, anche quello di non avere delle sedi idonee, però credo che davanti ad obiettivi di questa natura tutto possa essere superato. per la risposta del Sottosegretario; attendiamo con fiducia la presentazione all'opinione pubblica di tutto quello che si è fatto e soprattutto che la Città di Palermo, capoluogo di Regione, grande fonte di materiale, possa essere protagonista in questo processo.

con riferimento alle problematiche rappresentate dai senatori interroganti Vita, Garavaglia Mariapia, Rusconi e Marcucci, concernenti le fondazioni e gli istituti di cultura, si rappresenta che i contributi ai predetti organismi culturali hanno subìto, sin dal 2002, progressive decurtazioni a seguito delle diverse leggi finanziarie. Nel decorso anno, a fronte di una previsione di stanziamento di 12.953.000 euro sul capitolo 3671 da parte della legge finanziaria 2008 per i contributi alle istituzioni culturali previsti dalla legge n. 534 del 1996 (norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali), in realtà, al netto degli accantonamenti predisposti dal Ministero dell'economia e delle finanze, la somma disponibile è stata di 8.016.000 euro, di cui 7.062.000 euro in favore degli enti inseriti nella tabella triennale 2006-2008 prevista dall'articolo 1 della citata legge n. 534 e 953.000 euro in favore degli enti culturali non inseriti nella predetta tabella. Per quanto riguarda l'opportunità di destinare, in sede di ridistribuzione degli accantonamenti, la somma di 2 milioni di euro per gli interventi previsti dalla legge n. 534 del 1996, ed in particolare per gli istituti compresi nella tabella triennale, si sottolinea che gli accantonamenti sono stati disposti dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito delle manovre finanziarie per il contenimento della spesa pubblica. canto suo, attesa la necessità di rivolgere la massima attenzione alle fondazioni ed agli istituti culturali, ha comunque assicurato il massimo impegno per garantire loro il necessario sostegno. Già per l'anno 2008, infatti, è stata assegnata al settore un'integrazione di risorse pari a circa 517.000 euro, mentre un importo pari a complessivi 2 milioni di euro sarà destinato al medesimo fine all'interno del bilancio ministeriale per il 2009.

che mi pare abbia, forse con dolore, sottolineato la triste veridicità di questa interrogazione, che ha avuto una replica, piuttosto che nel merito, nelle competenze, nel senso che c'è un rinvio all'eventuale, del tutto eventuale, disponibilità del Ministero dell'economia. Sappiamo come funziona l'attività di questo Governo, c'è un superministero da cui altri discendono; mi preme però, in questa sede, evocare due questioni. La prima è che è noto al sottosegretario Giro e al ministro Bondi - l'attività culturale in Italia dovrebbe, in un Governo, per così dire, normale, essere in testa alle priorità, essendo l'Italia il Paese che è dotato di un patrimonio culturale primo al mondo.

allora questo Governo correggere la tendenza che porta alla distruzione sistematica di quasi tutto il lavoro culturale del Paese, dai beni culturali all'attività dello spettacolo, per non parlare poi - non è materia di questa interrogazione - della grande questione della formazione e della scuola? Infine, si sollevava, con i colleghi Garavaglia, Rusconi e Marcucci, un punto assai sentito dall'Associazione delle istituzioni di cultura italiane (AICI), che chiedono davvero poca cosa, e cioè di poter sopravvivere, non di più. È la richiesta di stare nella linea d'ombra di un galleggiamento difficile, trattandosi peraltro di istituzioni culturali che fanno dell'Italia un Paese di riferimento nel mondo. Si tratta di quelle istituzioni che divulgano il grande sapere italiano, la sua storia, la sua enciclopedia; quindi, la cifra ricordata di 517.000 euro non so

degli operatori, degli intellettuali, che forse indegnamente io qui sto rappresentando, di un Paese così straordinario: ripensateci! Diceva un grande economista, Claudio Napoleoni "Cercate ancora".

La realizzazione della «Nuova Romea» è un intervento ricompreso nel più ampio progetto Orte - Mestre di cui alla proposta presentata dal gruppo Gefip Holding S.A. più altri, promotore dell'intervento, e dichiarata di pubblico interesse da parte dell'ANAS. Avverso la dichiarazione di pubblico interesse deliberata dal consiglio di amministrazione di ANAS nel dicembre 2003 è stato proposto, da parte di un altro aspirante promotore, ricorso, accolto dal TAR del Lazio nella seduta del 18 giugno 2008. Contro la decisione del TAR è stato presentato, da parte di ANAS e del promotore, appello al Consiglio di Stato che nella riunione del 9 gennaio ultimo scorso ha rinviato l'esame del ricorso all'udienza del prossimo 3 marzo 2009. In merito allo stato di manutenzione e di sicurezza della statale 309 si rammenta che ANAS, da sempre attenta alle problematiche della sicurezza, si è impegnata ad investire oltre 28 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza della statale Romea, in gran parte aggiuntivi rispetto ai programmi stabiliti. Tale impegno, assunto con i rappresentanti degli enti locali, fa seguito ad un sopralluogo congiunto effettuato lo scorso 19 settembre. In tale occasione sono stati individuati interventi da attivare nel corso del 2009 per circa 12 milioni di euro, che riguarderanno la pavimentazione con asfalto ad alta aderenza, 1'installazione di nuove barriere di sicurezza, l'integrazione della segnaletica verticale anche con pannelli a messaggio variabile e l'installazione di puntuali sistemi di controllo della velocità. Entro il prossimo mese di febbraio 2009 verranno aggiudicate le gare relative alla manutenzione straordinaria delle pavimentazioni su tutta la statale 309 Romea, la segnaletica orizzontale in colato plastico nonché la fornitura e posa di nuove barriere sull'intera tratta della statale 309 e la statale 309-dir. Inoltre, entro il mese di marzo saranno aggiudicate le gare relative al progetto di implementazione della segnaletica verticale, complementare e pannelli a messaggio variabile sulle intere tratte delle due statali suddette. Sempre nel mese di marzo, sarà aggiudicato lo stralcio del progetto di messa in sicurezza della statale in questione, mediante la razionalizzazione delle intersezioni e la realizzazione di rotatorie e di piazzole di sosta in Provincia di Ravenna. invece in corso di definizione l'analogo progetto relativo al primo stralcio di messa in sicurezza della statale in Provincia di Ferrara, mediante la razionalizzazione delle intersezioni, la realizzazione di rotatorie e di piazzole di sosta riguardante la rotatoria di via dei Tigli a Lido degli Estensi e la razionalizzazione di altre intersezioni con viabilità provinciale. L'importo complessivo delle opere in fase di appalto lungo la statale 309 ammonta a euro 18.372.192,56. Il programma dei lavori è stato concordato dall'ANAS con la Regione Emilia-Romagna e le due Province di Ferrara e di Ravenna che, a loro volta, hanno coinvolto gli enti locali interessati. La Regione Emilia-Romagna e le due Province di Ferrara e di Ravenna hanno assicurato la massima collaborazione all'ANAS, anche in relazione all'acquisizione da parte dei Comuni delle aree necessarie per l'esecuzione dei lavori. ANAS conferma che il suo impegno, in accordo con le istituzioni locali, riguarda l'intero tracciato della Romea.

«Terraglio e Romea, strade killer». Infatti, dal momento in cui ho presentato questa interrogazione - era la fine del periodo estivo - ad oggi, su quella strada si è continuato a morire.

delle vacanze estive, quando il sovraffollamento dovuto al traffico turistico e al concentrarsi del traffico pesante ha comportato gravi lutti.

si tratta di capire, visto che il progetto non è ancora stato definito nella sua compiutezza, come si intenda procedere in contemporanea alla messa in sicurezza della statale Romea, soprattutto nel tratto Chioggia-Mestre, che è quello più devastato devastato e anche più pericoloso. Contemporaneamente, si prosegue l'opera di completamento del sistema infrastrutturale della Venezia Sud, che è colpita da incidenti per il sovraffollamento di mezzi pesanti, ma soprattutto rimane completamente assente dall'asse di sviluppo della infrastrutturazione.

di fare in modo che gli impegni illustrati ora dal Governo per la messa in sicurezza della strada siano davvero effettivi nei tempi e concordati con gli enti locali, gli enti locali, che l'opera di completamento della progettazione della Romea commerciale avvenga con il coinvolgimento degli enti locali interessati e che si completi il quadro infrastrutturale della Venezia Sud.

la statale Romea, da Chioggia a Mestre, è l'unica via di scorrimento per raggiungere Venezia, essendo stata abbandonata la via della comunicazione marittima. Eliminare dei sistemi di trasporto

con riferimento alla problematica denunciata dai senatori Lusi, Legnini, Rutelli e Marini, relativa alle condizioni di deterioramento dello storico ponte sul fiume Liri, bene di proprietà della Provincia dell'Aquila, si rappresenta che il Ministero, attraverso le proprie articolazioni periferiche (Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici per l'Abruzzo e Soprintendenza di settore), ha posto in essere le iniziative di propria competenza. Il giorno 25 agosto 2008 un architetto della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per l'Abruzzo, con sede a L'Aquila, ha effettuato un sopralluogo presso il citato ponte da cui è emerso che l'inadeguato stato di conservazione della struttura è stato determinato da mancata manutenzione. In particolare, i muri dei parapetti della sede stradale presentavano alcuni tratti privi, parzialmente, del paramento murario nonché della copertina di coronamento. Le attività di osservazione dello stato dei luoghi non hanno permesso, però, di stabilire con certezza se i danni rilevati siano stati generati da incuria ovvero da atti dolosi. Peraltro, anche le strutture portanti del ponte sono risultate a rischio di ulteriori danni a causa della vegetazione particolarmente rigogliosa ed incolta presente lungo gli argini del fiume. In virtù di quanto accertato ed in considerazione del fatto che il ponte, per le sue caratteristiche storiche ed artistiche, è ascrivibile fra i beni di rilevante interesse culturale ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio), la Soprintendenza, con lettera datata 4 settembre 2008, ha richiesto un intervento di urgenza alla Provincia de L'Aquila ed al Comune di Capistrello, sia a tutela dell'incolumità pubblica sia a salvaguardia del bene architettonico. L'amministrazione provinciale de L'Aquila, in data 17 ottobre 2008, ha comunicato alla Soprintendenza che i lavori di ripristino del parapetto del ponte verranno eseguiti con le risorse del corrente anno. Nel frattempo, ha provveduto a ripristinare le condizioni di sicurezza e ad evitare ulteriore sottrazione illecita di materiale, ponendo in essere alcuni interventi quali l'asportazione delle copertine in pietra distaccate ed il loro stoccaggio presso i magazzini della Provincia, nonché l'installazione provvisoria di paletti in legno e rete in plastica lungo i parapetti.

le due basi verticali murarie delle pietre lapidee, ahimè a valle dell'asportazione delle stesse, come lei sa da interrogazione depositata e, soprattutto, da verbale, credo, delle forze dell'ordine intervenute sul luogo.

diventa oggetto di attenzione ed obiettivo di intervento da parte delle strutture competenti dello Stato e degli enti locali e territoriali

invitando le amministrazioni competenti ad intervenire proprio su quella vegetazione rigogliosa e incolta, che è una delle cause delle cause della cattiva manutenzione del ponte, ma che non riguarda la questione dell'asportazione delle pietre lapidee. Dal momento che le pietre insistono su quel ponte, è evidente che un intervento alla struttura del ponte stesso è anch'esso è anch'esso necessario e urgente per realizzare il doppio fine: se da una parte non vengono rubate, perché oggi quelle residue sono state asportate per essere stoccate nei magazzini della Provincia, che dovranno poi provvedere con fondi propri - questa è una notizia che registriamo oggi e la ringrazio, Sottosegretario ad un intervento manutentivo, dall'altra, si deve fare in modo che quando questo intervento sarà terminato non ci sia un problema legato alla struttura stessa del ponte, che peraltro è l'unico mezzo di collegamento tra la Valle del Liri, in Abruzzo, e la Regione Lazio.

il collegamento ferroviario sulla linea Roma-Pescara è compreso nei servizi di interesse regionale regolati, in quanto tali, con contratto di servizio stipulato dalla Regione ai sensi del decreto legislativo n. Tali servizi esulano, pertanto, dalle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al fine di fornire comunque un adeguato riscontro alla richiesta di notizie avanzata dall'interrogante, è stata sentita la società Ferrovie dello Stato che ha quindi riferito quanto segue. La tratta Roma-Pescara è oggetto di una serie di interventi di potenziamento e velocizzazione in parte già attivati, in parte in progettazione. A ottobre 2006, è stato attivato il nuovo tratto indipendente di accesso nel nodo di Roma della linea Alta Velocità/Alta Capacità (AV/AC) Roma-Napoli che ha consentito di eliminare le interferenze dei treni AV/AC sul traffico della tratta Roma-Pescara tra Prenestina e Salone. A luglio 2007, è stato attivato il tratto di raddoppio tra Salone e Lunghezza e, a maggio 2008, è stato attivato l'attestamento a Lunghezza dei treni della linea Roma-Guidonia. Per quanto riguarda, quindi, il potenziamento infrastrutturale della linea, si rappresenta quanto segue. Relativamente al raddoppio della linea tra Lunghezza e Guidonia, ad agosto 2008 sono stati trasmessi al Ministero delle infrastrutture gli elaborati di progetto per la riapertura della conferenza di servizi, la cui data non è stata ancora fissata. Questo nuovo tratto a doppio binario, incrementando la capacità del segmento di linea più carico di traffico, consentirà di potenziare progressivamente il servizio regionale su tale asse. Il CIPE, con delibera n. 85 del 29 settembre 2002, ha impegnato RFI a sviluppare lo studio di fattibilità di sette collegamenti ferroviari nel Mezzogiorno d'Italia, tra i quali quello tra Roma-Pescara. Lo studio di fattibilità redatto ha proposto uno scenario infrastrutturale finalizzato a rendere competitivo il sistema ferroviario rispetto alle altre modalità di trasporto e a garantire migliori livelli prestazionali dell'offerta in termini di tempi di percorrenza. Il CIPE con delibera n. 91 del 2004 ha approvato tale studio di fattibilità che ha individuato interventi di velocizzazione, consistenti essenzialmente in tratti di raddoppio e varianti plano-altimetriche, dell'importo stimato in circa 1.184 milioni di euro. II contratto di programma 2007-2011 tra RFI e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il potenziamento della linea Roma-Pescara prevede: la realizzazione del raddoppio Lunghezza-Guidonia, in tabella A «Opere in corso», con un costo di 102 milioni di euro, valutato sulla base della progettazione definitiva sviluppata; la progettazione dell'intervento «Roma-Pescara», in tabella A, con un costo di un milione di euro, del quale, ai sensi della citata delibera del CIPE n. 85 del 2002 è stato sviluppato lo studio di fattibilità; la realizzazione degli interventi di cui al progetto «Roma-Pescara», in tabella C «Altre opere da realizzare», con un costo stimato di 1.184 milioni di euro. A marzo 2008, RFI spa, in relazione a quanto approvato dal CIPE con delibera n. 91 del 2004, ha inoltrato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il progetto preliminare «Velocizzazione della linea Roma-Pescara», per l'attivazione dell'istruttoria necessaria all'avvio dell'*iter* approvativo da parte del CIPE. Il progetto presentato riguarda la realizzazione di cinque varianti da realizzare prioritariamente, consistenti nel: raddoppio "Tivoli", da Guidonia a Vicovaro; raddoppio Celano-Bugnara; variante "Pratola" che permette di eliminare le tortuosità di tracciato fra Sulmona e Pratola Peligna, con dismissione della linea attuale; variante "Manoppello", a singolo binario, che consente di bypassare i centri abitati di Brecciarolo, Manoppello e Manoppello Scalo e di collegare il nuovo interporto di Val Pescara in fase di realizzazione. Il progetto prevede, inoltre, la realizzazione della nuova fermata di Manoppello Scalo e la dismissione della linea esistente. linea Chieti-Pescara. L'investimento di tutti gli interventi ammonta a oltre 1.550 milioni di euro, con tempi di realizzazione di poco inferiori a otto anni. Il progetto preliminare sviluppato ha riguardato anche altri interventi, per un investimento complessivo di ulteriori 1.400 milioni di euro, finalizzati al completamento della velocizzazione della linea, che saranno realizzati progressivamente secondo le disponibilità finanziarie. Tali interventi consistono nella realizzazione di un ulteriore tratto di raddoppio fra Vicovaro e Tagliacozzo e delle due ulteriori varianti "Popoli" e "Scafa". Si sottolinea, infine, che la disponibilità dei soli 168 milioni di euro, citati dall'interrogante, non permetterebbe di realizzare alcun intervento significativo, neanche il solo raddoppio di "Tivoli" da Guidonia a Vicovaro, il cui costo, sulla base del progetto preliminare sviluppato, è stato stimato pari a circa 330 milioni di euro. Per quanto riguarda, infine, l'attestamento dei treni provenienti da Pescara nella stazione di Roma Tiburtina, si evidenzia che l'assetto regolatorio del nodo di Roma, realizzato in ottica di massimizzazione della capacità degli impianti ed in particolare di Roma Termini, prevede che la linea proveniente da Pescara-Sulmona abbia il naturale attestamento nella stazione di Roma Tiburtina, al fine di separare i flussi di traffico provenienti dalla linea Alta velocità Napoli-Roma da quelli provenienti dalla citata linea Sulmona-Pescara. In deroga all'assetto regolatore del nodo, che, come sopra detto, prevede la separazione dei flussi di traffico Alta velocità con quelli della linea da Pescara, per tenere conto delle sollecitazioni dei pendolari della linea da Sulmona che richiedevano la conferma su Roma Termini dei citati quattro treni pendolari, si è autorizzato l'arrivo a Roma Termini del solo treno 2371 Sulmona-Roma che rappresentava la richiesta prioritaria dei pendolari. Per quanto riguarda i tempi di percorrenza, si sottolinea il fatto che, contestualmente all'attivazione del doppio binario da Salone a Lunghezza, l'offerta sulla relazione metropolitana Lunghezza-Roma è stata significativamente incrementata, passando da un servizio orario a un servizio ogni 30 minuti, con rinforzi nelle fasce di punta. In ogni caso, nella tratta metropolitana, le tracce orarie dei servizi regionali provenienti da Sulmona-Pescara devono necessariamente armonizzarsi con i servizi metropolitani

Come avrete avuto modo di leggere, lei e gli uffici che l'hanno aiutata nell'istruzione di questo argomento, nell'interrogazione ci sono precise e puntuali proposte con domande abbastanza chiare. Inoltre, il sottoscritto, come gli Uffici del Senato hanno dimostrato attraverso telegrammi inviati ai Ministeri competenti con una puntualità certosina, consegnati anche al sottoscritto per conoscenza, ha insistito con i Ministeri competenti perché si rispondesse ogni volta che in Aula si sollecitava questo tipo di risposta. Ora, lei, signor Sottosegretario, a nome del Governo, ci viene a dire che che praticamente è tutto o quasi a posto, nel senso che ci ha fornito una notevole illustrazione di opere da realizzare, decise con una lentezza stratosferica (mi rivolgo ad una persona che so essere efficiente, non solo per la sua provenienza, ma anche per la sua storia personale). a dirci che uno studio di fattibilità, approvato nel 2004, richiesto nel 2002, oggi vede una cifra di 1.184 milioni di euro previsti e mai finanziati; che nel marzo 2008 sono stati decisi progetti di interventi per 1.550 milioni di euro, decisi e mai finanziati; che gli unici soldi che questo Parlamento ha stanziato dal 1997 ad oggi sono 168 milioni, non non per fare i quattro raddoppi e l'intervento di collegamento con il porto di Pescara che lei ci ha descritto oggi (che non servono assolutamente a niente, né ai pendolari né a quelli che usufruiscono di quella linea ferroviaria). Ci ha comunicato che proprio quei soldi, come ho detto gli unici stanziati, in realtà non servono a realizzare le opere di ammodernamento necessarie per la funzionalità di quella linea ferroviaria.

messo nel tempo di percorrenza di questa linea ferroviaria è tale per cui il treno, per rispettare i larghi spazi indicati da Ferrovie, si deve fermare in alcune stazioni 8, 10 o 12 minuti solo per rispettare quel tempo; e perché? Perché, come lei ha detto correttamente all'inizio della sua risposta, quella è una tratta ferroviaria soggetta ad un contratto di servizio tra Ferrovie dello Stato e Regione competente per territorio (quindi, per una parte, Regione Abruzzo e, per l'altra parte, Regione Lazio), e in tal modo Ferrovie non doveva pagare le penalità derivanti dai ritardi. Così i pendolari impiegano un tempo infinito per spostarsi dai loro comuni di residenza fino ai luoghi di lavoro, sottostando a ritardi incredibili, perché l'organizzazione del tempo di percorrenza è tale per cui - come dicono i ferrovieri competenti, le organizzazioni sindacali e i dirigenti di Trenitalia e di RFI che

Aspettate a rispondere ancora di più perché, guarda caso, nella Regione principalmente interessata da quella tratta, c'è una elezione straordinaria del Consiglio regionale e c'è un signor Presidente del Consiglio che va a promettere 19 miliardi di euro per per realizzare opere infrastrutturali, indicando chiaramente, in più luoghi di quella Regione Abruzzo, il raddoppio della linea ferroviaria quando nessuno gliel'aveva mai chiesto. Ma cinque mesi prima, nel primo decreto-legge che avete approvato in Consiglio dei ministri, avete cancellato i 168 milioni di euro necessari necessari per realizzare gli investimenti infrastrutturali in quella Regione, gli unici investimenti dal 1997 in poi - quindi tutti i Governi che hanno preceduto il vostro sono corresponsabili - e assolutamente necessari per realizzare interventi strutturali in quella Regione.

questa interrogazione, insieme ai cittadini che, stressati come sono, si rivolgono a voi, a noi, alla politica, al Parlamento e all'azienda interessata per analizzare i problemi, la invitiamo a valutare che gli interventi che voi proponete con i quattro raddoppi non servono a nulla, tranne il primo, corretto, che è l'intersezione, come lei ha spiegato molto bene,

interventi di ammodernamento dei meccanismi di funzionamento della tratta, nient'altro: non servono cifre faraoniche che comportino appalti che non si realizzeranno mai. Lei è stato onesto intellettualmente e politicamente nel dire che ci vogliono otto anni per realizzare quegli interventi, ma lei sa, per la sua esperienza, maggiore della mia, che non ne non ne basteranno 16 e nemmeno 24 di anni, perché è una di quelle opere classificate, indipendentemente dalla tabella, come di serie C quanto ad importanza e, quindi, non sarà mai necessaria. È evidente che se continuerete a trattare i cittadini in questo modo, i cittadini sapranno con chi prendersela. Almeno Senatore Lusi, per correttezza di informazione e non per difendere il sottosegretario

II sistema Sarmento-Monte Cotugno è costituito da un invaso di circa 530 milioni di metri cubi realizzato sul fiume Sinni mediante uno sbarramento in terra di 65,5 metri di altezza da tempo realizzato nel quale, tramite adduttore idraulico, dovranno inoltre confluire le risorse idriche captate dalla traversa sul fiume Sarmento ubicata nel Comune di San Giorgio Lucano (con un bacino sotteso di circa 175 chilometri quadrati). L'intero sistema viene gestito, anche in fase di realizzazione delle rimanenti opere, dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia, Basilicata ed Irpinia I lavori relativi alla traversa sono stati ultimati, ma non è stata ancora raggiunta la piena funzionalità del sistema, poiché la realizzazione dell'adduttore idraulico, prevista mediante una galleria a pelo libero della lunghezza di circa 4.570 metri, ha subìto nell'anno 2005 un'interruzione dei lavori per difficoltà tecniche intervenute durante l'esecuzione, quando mancavano circa 400 metri al completamento dell'opera di perforazione, oltre al rivestimento definitivo di circa 1.560 metri. In particolare, durante i lavori si registravano fuoriuscite dal fronte di scavo di materiale fluido composto da acqua in pressione frammista a materiale limo-sabbioso con inondazione progressiva di un tratto di galleria di 200 metri. Ciò ha determinato l'instaurarsi di un contenzioso con l'impresa appaltatrice dei lavori, terminato nello scorso mese di giugno 2008 con la rescissione del contratto e l'affidamento da parte dell'EIPLI dei rimanenti lavori ad una nuova impresa per l'importo di circa 6.800.000 euro. L'originario intervento di completamento della condotta idrica Sarmento-Monte Cotugno, si ricorda, era stato finanziato, d'accordo con la Regione Basilicata, dal Ministero dei lavori pubblici nell'ambito del cofinanziamento europeo di cui al programma operativo «risorse idriche», per un importo di 18.442.955,24 L'opera, tuttavia, non poteva essere completata dall'ente attuatore nel termine del 31 dicembre 2001 tassativamente stabilito dalla normativa del programma di finanziamento comunitario. Non di meno il Ministero il Ministero ottenne dalle autorità comunitarie che per questo, come per altri analoghi interventi, non occorresse il definanziamento, a fronte dell'impegno al completamento degli stessi nell'ambito del successivo periodo di programmazione 2000-2006. Con apposito protocollo d'intesa tra il Ministero e la Regione Basilicata in data 17 febbraio 2005, veniva convenuto che in particolare le rimanenti opere di completamento dell'intervento in questione avrebbero fatto integralmente carico al Programma operativo regionale (POR) gestito dalla stessa Regione Basilicata. Tuttavia, il Ministero, in qualità di soggetto competente per la stipula degli accordi di programma interregionali per il trasferimento di risorse idriche previsti dall'articolo 17 della legge n. 36 del 1994 (la cosiddetta legge Galli), come modificato dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 152 del 2006, vigila con attenzione 1'andamento del completamento dell'opera. Infatti, la realizzazione della condotta idrica Sarmento-Monte Cotugno, parte integrante del sistema idrico ionico Sinni, consentirebbe di liberare risorse fino a circa 35-40 milioni di metri cubi d'acqua in favore della Puglia, come già previsto nell'accordo di programma stipulato tra le Regioni Basilicata e Puglia e l'allora Ministero dei lavori pubblici nel 1999. Di riflesso ciò permetterebbe presumibilmente di rendere fruibili alcune opere attualmente inutilizzate costituenti il sistema di irrigazione del Salento (invaso del Pappadai, acquedotto del Sinni irriguo), rendendo finalmente produttivi i circa 267,21 milioni di euro non attualizzati finanziati dal 1980 dallo Stato e contribuirebbe alla riduzione del prelievo da falda nella penisola salentina. Da informazioni apprese da fonti del soggetto gestore della realizzazione dell'opera, il già citato EIPLI, i lavori, consegnati sotto riserva di legge all'impresa affidataria in data 1° agosto 2008, sono nella fase preliminare di installazione del cantiere e di esecuzione delle indagini propedeutiche alla definizione del dettaglio esecutivo delle lavorazioni idonee alla ripresa dello scavo. Sebbene la data prevista di ultimazione dei lavori del 31 luglio 2009 presumibilmente non essere rispettata, sarà cura dell'Amministrazione vigilare affinché i lavori procedano con la necessaria celerità.

questioni sollevate nell'interrogazione e soprattutto per l'impegno, che è stato ribadito, di vigilanza da parte del Ministero su quest'opera.

è oggetto di lavori di adeguamento della sezione stradale al tipo III delle norme C.N.R. 80, attualmente in corso di esecuzione, e concerne i lotti 8 e 9. Relativamente al lotto 8, tra le progressive chilometriche 432-890 e 444-653, dallo scorso 8 agosto la sede stradale è interamente percorribile nelle due direzioni a doppio senso di marcia. Il lotto 9, tra le progressive chilometriche 444-653 e lo svincolo per Metaponto, risulta percorribile a doppio senso di marcia per entrambe le direzioni mentre persiste, in corrispondenza dello svincolo di Metaponto, un'ampia rotatoria provvisoria a doppio senso di marcia. Durante i fine settimana e nelle ore di più intenso transito veicolare, d'intesa con la polizia stradale, l'ANAS ha istituito un presidio per la regolamentazione del traffico.

che ha voluto fornire per quanto riguarda la gestione dei punti di crisi del traffico veicolare, colgo l'occasione per pregarla di seguire tempestivamente il completamento di questa arteria che potrebbe dare un contributo straordinario